L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868,

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e nella mia responsabilità di Presidente della Commissione giustizia, che non è dissimile dalla responsabilità che, comunque, riguarda anche la Presidenza del Senato. Sotto questo profilo, mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore, senatore D'Ascola, e del vice ministro Costa.

nel corso dell'ultima seduta è stato respinto un emendamento del senatore Barani che prevedeva un aumento di pena per il reato di concussione commesso da un appartenente all'ordine giudiziario. Ciò detto, signor Presidente, desidero segnalare una palese incostituzionalità nel testo che stiamo andando ad approvare, con con la conseguenza di mettere le basi per una navetta tra la Camera ed il Senato e, quindi, sostanzialmente, di ritardare l'approvazione del disegno di legge in tema di corruzione che tanto a cuore sta, oltre che alle forze politiche, anche al Paese. Il tema è abbastanza semplice. A seguito della votazione dell'articolo 1

Questa pena è superiore sia alla pena per il reato di concussione per induzione (che va da sei a dieci anni e sei mesi), sia alla pena per concussione, che va da sei a dodici anni, il che equivale a dire che il reato di corruzione in atti giudiziari viene ad essere punito in maniera più grave identica al reato di concussione commesso da un appartenente all'ordine giudiziario. Questo evidentemente, sotto il profilo della ragionevolezza, espone questo provvedimento ad una censura di incostituzionalità, perché essendo pacifica la maggiore gravità del reato di concussione rispetto al reato di corruzione, non c'è davvero nessuna ragionevolezza nell'immaginare che il reato di corruzione commesso da un magistrato venga punito in misura maggiore o uguale rispetto al reato di concussione commesso dallo stesso magistrato. È vero che un disallineamento delle sanzioni vi era anche prima, cioè con la legge Severino, perché il reato di corruzione in atti giudiziari era punito in termini maggiori rispetto al reato per concussione per induzione, ma questo poteva trovare una giustificazione nell'affermare che il legislatore riteneva il reato di corruzione in atti giudiziari più grave del reato di concussione semplice commesso da un pubblico ufficiale qualunque. Nel momento, però, in cui si aumentano le pene nel modo in cui le abbiamo aumentate e ci troviamo di fronte ad un'ipotesi non prevista dalla legge Severino, e cioè che la corruzione in atti giudiziari è punita in termini identici alla concussione per costrizione, irragionevolezza della sanzione è lampante. Sotto questo profilo credo quindi, ove mai il Governo intenda evitare la navetta tra Camera e Senato, ovvero intenda evitare di esporre la presente norma al giudizio della Corte costituzionale, che sarà inevitabilmente di illegittimità costituzionale, che vi sia ancora tempo per il Governo e per il relatore di presentare un emendamento che individui il reato di concussione in atti giudiziari e sostanzialmente in questo modo venga a sanare una palese illegittimità costituzionale. Questo emendamento non sarebbe precluso

rispetto al reato di concussione, immaginando un emendamento che configuri la concussione in atti giudiziari si immaginerebbe una figura autonoma di reato che, una volta adeguata la sanzione alle sanzioni previste nel reato di corruzione in atti giudiziari, sanerebbe completamente la questione. Era mio dovere rappresentare all'Assemblea,

evidente che, nel momento in cui si dovesse cambiare la norma alla Camera, vi sarebbe una navetta la cui responsabilità, con riferimento alla lunghezza dei tempi, non può che assumersi il Governo, ovvero, ove questa navetta non ci dovesse essere e dovesse esservi il giudizio di illegittimità della Corte costituzionale, di questo giudizio di illegittimità non potrebbe che farsene carico il Governo, essendo stata la questione chiaramente denunciata in Aula nel corso dei lavori.

Palma, invito il relatore e il vice Ministro a tenere presente questa osservazione, perché il mio Gruppo e le opposizioni ovviamente facciamo opposizione sul merito, ma di fronte a una lapalissiana incongruenza costituzionale - la Costituzione, ripeto, è stata fatta dai nostri Padri costituenti che volevano

Per non essere accusati di ostruzionismo, noi stiamo dando una mano al Governo e al Paese, anche se dissento dal presidente Palma, perché non credo proprio che

Il testo originario prevedeva che la somma da pagarsi a titolo di riparazione la si potesse disporre non soltanto con la sentenza di condanna pronunciata in un giudizio ordinario, ma anche con la sentenza di condanna pronunciata a seguito di patteggiamento. emendamento propone l'eliminazione di quest'ultimo riferimento, ossia la possibilità di imporre l'obbligo della riparazione soltanto con la sentenza penale di condanna e non anche con la condanna pronunciata a seguito di patteggiamento.

che prevedeva la possibilità di ordinare la riparazione, vuoi con la sentenza di condanna, vuoi con la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento, non si confrontava ancora con l'emendamento governativo introdotto all'articolo 5, ossia quello che prevede quale ragione per l'ammissione al patteggiamento l'obbligo di restituire il provento illecito a carico dell'indagato il quale chiede di patteggiare. il relatore si è posto il problema della convergenza tra questo obbligo, che costituisce un vero e proprio presupposto per la possibilità di chiedere il patteggiamento chiunque intenderà patteggiare saprà in anticipo che questa possibilità risulterà condizionata alla restituzione), e la somma da pagarsi a titolo di riparazione, che era prevista originariamente nel testo dell'articolo 3. Non c'era però soltanto questo aspetto

si prevede, non soltanto l'obbligo di ordinare la restituzione, ma anche di disporre la riparazione a carico del condannato a favore dell'amministrazione di appartenenza

che frequentemente si intreccia con quello del patteggiamento tutte le volte in cui chi intende patteggiare la condanna chiede anche che la stessa sia condizionalmente sospesa.

più disposizioni dotate del medesimo contenuto precettivo. La necessità è ovviamente quella di determinare un qualche ordine e una qualche razionalità per evitare l'affollarsi di istituti analoghi sulla stessa fattispecie. C'è poi da dire - e qui il relatore conclude il suo intervento - che abbiamo avvertito la necessità di disallineare la condanna pronunciata a seguito di giudizio ordinario rispetto alla condanna pronunciata nell'ambito del patteggiamento.

Lo Stato ha interesse al patteggiamento tutte le volte in cui ovviamente ne ricorrano le condizioni, tra le quali oggi sappiamo che c'è anche l'obbligo della restituzione. Stabilire le stesse conseguenze sanzionatorie per il caso di una sentenza di condanna pronunciata dopo un lungo giudizio e di una sentenza di condanna pronunciata dopo il semplice patteggiamento avrebbe determinato l'evidente conseguenza che nessuno avrebbe patteggiato e tutti avrebbero preferito la soluzione costituita dal giudizio ordinario.

affermare di aver riscontrato non meglio identificati errori nella denuncia presentata dai singoli contribuenti, di solito per cifre modeste che molti contribuenti ritengono di sanare pagando piuttosto che perdere tempo ad andare a raccogliere la documentazione, prendere l'appuntamento con l'Agenzia delle entrate, parlare con un dirigente, sperando di trovarlo

cerca di non pagare anche ciò che sarebbe dovuto e pertanto andrebbe sanzionato, mentre il cittadino colpito da queste richieste andrebbe modestamente risarcito. Io sono stato attento nel porre la sanzione

della Commissione bilancio, che invece avrebbe dovuto esprimere un parere particolarmente favorevole perché alla fine, siccome al responsabile della richiesta indebita di pagamento si chiede 100 e a colui che è stato colpito si dà 80 (fatte salve alcune spese), c'erano ampiamente i margini perché lo Stato incassasse ancora

non si dovessero più fare richieste indebite di pagamento lo Stato ci perderebbe troppo; tuttavia, se lo Stato campa con le richieste di pagamento ingiuste, allora abbiamo qualche problema che va ben al di là dell'articolo 81 della ad incidere sui diritti fondamentali della Costituzione, che sono perfino più importanti del rispettatissimo articolo 81, talmente rispettato che dopo 70 anni di applicazione abbiamo 2.000 miliardi di debiti.

tra l'altro, è stato sollevato un dubbio di costituzionalità su quanto stiamo per andare a votare, se riuscissimo ad avere una risposta dal relatore e dal Governo. Altrimenti, delle due l'una: o non sanno cosa rispondere o forse non è arrivato il verbo di Palazzo Chigi.

siamo stati direttamente chiamati a dare una risposta, relatore e Governo, e la risposta c'è. Ovviamente, il problema posto dal Presidente della Commissione giustizia è un problema noto; ma è un problema noto prima e a prescindere da questa riforma. Sappiamo bene che che il delitto di corruzione in atti giudiziari esiste non certo da oggi e che il delitto di concussione è un delitto di tipo generalista. Ossia,

che appartiene all'ordine giudiziario. Già basterebbe questa risposta. Non è un problema nuovo, ma un problema già esistente. Peraltro, c'è da dire che non ci troviamo in una situazione di squilibrio sanzionatorio, ma di perfetto equilibrio sanzionatorio. Il Presidente della Commissione giustizia sostiene che in questo contesto si potrebbe individuare uno squilibrio, perché la concussione eventualmente operata

parlo anche della riforma del 2012, alla quale gli stessi parlamentari che oggi pure si dolgono hanno partecipato.

sia stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale. Questo non vuol dire che non possa essere proposta ora, ma che si tratta di un problema esistente.

un pubblico ministero, ovvero da un giudice e, quindi, più riassuntivamente, da un appartenente all'ordine giudiziario, questi fatti dovrebbero essere puniti diversamente.

quell'emendamento sarebbe stato accolto. Tra l'altro, è una materia che avrebbe implicato una meditazione diversa. Ad esempio, come si costruisce questa concussione del magistrato? Nelle forme duplici della concussione per costrizione? Della concussione attenuata: l'indebita induzione? Si costruisce con le aggravanti del capoverso del delitto di corruzione in atti giudiziari? Insomma, il dibattito su questo punto non è stato neanche stimolato nell'ambito delle discussioni e, quindi, era certamente un dibattito immaturo. Nulla vieta, a coloro i quali intenderanno sollevare la questione, di porre un'espressa questione, proponendo però un testo che si faccia carico di tutti problemi dei quali questo testo certamente non si era fatto carico.

Presidente, ho apprezzato la bravura del relatore nel tentare di giustificare qualche cosa che giustificabile non è. Nel 2012, quelli di noi che erano in quest'Aula con me, hanno votato la legge anticorruzione con aumenti di pena, ma si manteneva l'equilibrio tra i vari reati. Che cosa è avvenuto? Che oggi non c'è più un equilibrio: la concussione viene punita meno gravemente della corruzione, sia pure della corruzione in atti giudiziari.

prima di determinare uno sconquasso che sarebbe peggiore dell'attuale situazione! Immaginate quale potrebbe essere lo scenario se, di fronte ad eventuali procedimenti, fosse sollevata

l'allungamento dei tempi dei processi di corruzione e probabilmente comporterebbe anche influenze su quella prescrizione cui tutti teniamo. Mi rendo conto c'è una risposta evasiva, ma nello stesso tempo dovrebbe essere preoccupazione di tutti di rendere queste norme concretamente applicabili e non farne solo uno *spot*!

il presupposto del ragionamento era che siccome all'articolo 5 è stato formulata una figura di patteggiamento diversa

sulle associazioni di tipo mafioso sono stato autore di alcune modifiche della normativa nella sia sotto il profilo delle pene, sia sotto il profilo di una migliore riscrittura delle norme che riguardano l'utilizzo del 41-*bis* e di altre norme che servono ad assicurare una vera lotta alla mafia.

ventiquattro anni il massimo della pena della reclusione. Per chi non lo ricordasse, per quelli come me che hanno sostenuto per anni

Inoltre, attraverso gli emendamenti 4.300, 4.302 e 4.305, formulo una rimodulazione degli aumenti in modo tale che vi sia coerenza e si arrivi con il massimo della pena a ventiquattro anni. Per tale ragione, vorrei che tutti, indipendentemente dall'appartenenza ai Gruppi di Forza Italia o del Partito Democratico, facessero un minimo di riflessione e di controllo su quello che ho detto, con il codice penale davanti. In questo caso, credo che un minimo di attenzione dovrebbe portare all'approvazione dei miei emendamenti. *(Applausi del

Pur comprendendo le difficoltà che presenta questo testo normativo per quanto riguarda un esame complessivo e l'assetto sistematico dell'introduzione delle norme, abbiamo ritenuto, in particolare riguardo all'articolo 4 (che prevede una modifica al reato di associazione di tipo mafioso, anche straniera), di proporre degli emendamenti volti sostanzialmente a prevedere un aumento di pena.

sanzione prevista per il famoso articolo 416-*ter* che, come ricordiamo tutti, è stato oggetto di esame del Parlamento lo scorso anno con un esito che ci ha visto contrari con la notoria, ricordiamolo, riduzione delle pene previste per il reato di scambio elettorale politico-mafioso del 42 per cento. Noi valutammo anche la quantità di pena ridotta con quel provvedimento. Quella misura fu giustificata (dalla maggioranza e, se ben ricordo, anche da parte dell'opposizione che siede alla nostra sinistra) sulla base di un principio: la necessità dell'asimmetria della pena tra il 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) e il 416-*ter* il testo che ci apprestiamo a votare prevede, tra le varie misure che aumentano le sanzioni, come è noto, anche l'aumento delle sanzioni per l'articolo 416-*bis*, la cui pena per la mera partecipazione è

sostanziale ed effettiva tra le pene edittali. Veramente non vediamo per quale motivo il Parlamento debba sottrarsi a questa possibilità di ripristinare una sanzione per l'odioso voto di scambio politico-mafioso secondo i criteri che sono anche rispettosi della logica che dalle altre forze politiche veniva sollevata per giustificare quella riduzione.

recente ha conosciuto una sua particolare accentuazione e una sua irresistibile pervasività, a una sorta di illusione punitiva affidata pressoché interamente all'innalzamento delle pene

che qualifica molti provvedimenti approvati in questa legislatura, sembra rispondere ad esigenze diverse da quelle della efficacia nella lotta contro la corruzione.

quanto testé ha affermato il senatore Manconi. Per dirla alla dantesca, non si perda ogni speranza entrando qui e sentendo che esiste anche una voce fuori dal coro di allineati, che fa una diagnosi, un esame obiettivo e una prognosi inconfutabili. Il senatore Manconi ha parlato di scientificamente provato, i massimi esperti della materia dicono che innalzare le pene *sic et simpliciter* non serve a nulla, è deleterio; quindi, ci stiamo massacrando, ci stiamo fustigando. Per cosa? Per fare piacere a chi? Per andare dove? Il senatore Manconi chiedeva dove fosse la prevenzione. Non esiste, questa grande sconosciuta.

dovere. Stiamo entrando in uno Stato che non è di polizia ma giudiziario, e noi sappiamo dalla storia che i regimi giudiziari, ovviamente giustizialisti, sono stati i peggiori che ha avuto il nostro Paese. In questo momento ne stiamo vivendo uno

L'incremento delle pene, anche se non mi aspetto che avrà un'immediata ripercussione sulla frequenza con cui i reati di cui stiamo parlando verranno perpetrati, segnala comunque una netta valutazione politica di questo Parlamento e una valutazione culturale nel Paese di riprovazione per questo genere di reati. Voglio ricordare ai colleghi che quando si parla di prevenzione, questi sono reati tipici della classe dirigente, ovvero reati di quelle persone che in qualche modo dovrebbero costituire dovrebbero costituire guida morale per il Paese e la cui mancanza di inclinazione in questo senso ha portato questo Paese alle condizioni in cui si trova adesso. Per questo motivo io e la componente che rappresento nel Gruppo Misto, Italia Lavori

Abbiamo trattato fino ad ora i reati di corruzione. Nell'articolo 4 è previsto l'aumento delle pene per il 416*-bis*, che - ripeto - punisce il reato di associazione mafiosa diretta; passeremo successivamente ad un terzo pilastro di questo disegno di legge, che è il falso in bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 416-*bis*, noi ci troviamo in questa condizione, colleghi: adesso i capi mafia,

stanno provando ad organizzarsi facendo in modo che questa parte, dove sono previste dalle pene pesantissime, sia appannaggio della cosiddetta manovalanza, per riservarsi quella parte che è di guida dell'associazione, intorno a cui sanno che le pene non sono così severe come per i reati fine. Ci troviamo pertanto nella condizione, che ci è stata segnalata anche in Commissione antimafia, su tutti i territori per cui, per scarcerazione per fine pena, abbiamo pericolosissimi *boss* che, appena ritornano fuori, immediatamente riprendono in mano la guida dell'organizzazione, diventando - questi sì - una minaccia per la democrazia, questi sì una minaccia letale per la dignità della persona e, in molti casi, anche per lo sviluppo economico di molti territori. Ecco perché la proposta che adesso ci apprestiamo a votare, che è contenuta nell'articolo 4, dà una risposta avanzata a questa evoluzione dell'organizzazione mafiosa, impedendo che, come democrazia, noi ci troviamo sotto minaccia da parte dei *boss* mafiosi e facendo in modo che a questa evoluzione strategica ed organizzativa lo Stato risponda per tempo, passando da quella «antimafia del giorno dopo» (che è stata sempre affannosa e sempre priva di respiro) ad un'«antimafia del giorno prima», che sia in grado di poter colpire quell'evoluzione facendo in modo che la democrazia prevalga sull'organizzazione mafiosa.

Dopo aver richiamato ripetute volte l'Assemblea a prestare attenzione al fatto che qua si sta votando il reato di associazione mafiosa e, così, sostanzialmente, sotto il profilo della suggestione, consigliarle qualsivoglia tipo di aumento di pena, alla fine il discorso del senatore Lumia si conclude e si risolve in due piccole circostanze. è quella di aver saputo, girando per i territori, di una certa attuale prassi dell'associazione mafiosa. Devo dire la verità: questa è la prima volta che il Parlamento legifera e modifica la norma su dei «sentito dire», senza dei controlli in ordine alla realtà giudiziaria di questo Paese. La seconda è che, sostanzialmente, i capi della mafia avrebbero la "furbizia" di non macchiarsi le mani dei reati di sangue o dei reati più gravi, così da poter scampare le relative sanzioni. Dicevo che ero e sono stupito. Vedete, noi possiamo aumentare le pene come meglio vogliamo, per cui, forse, potevate aderire ad un emendamento del senatore Giarrusso che, seguendo forse lo stesso ragionamento del senatore Lumia, reclamava per i capi di un'associazione mafiosa armata la pena dell'ergastolo e così avremmo chiuso tutti quanti i giochi. Ma, nella realtà, ci troviamo di fronte ad un reato di pericolo. Quindi non vi è un danno, non vi è una lesione effettiva di un interesse, salvo quella propria del reato di pericolo, che è l'ordine pubblico. Prendiamo atto, allora, che il reato è di particolare gravità, ma non riusciamo a comprendere in che modo questa forsennata corsa agli inasprimenti sanzionatori possa trovare soddisfazione, in ciò denunciando il suo essere squisitamente propagandistico, nell'affermare che la pena da sette

che denunciano esclusivamente la manovra propagandistica che è alla base di questo provvedimento. Ma tant'è, lo si vuole fare e lo si faccia. Ma dove davvero rimango stupefatto è quando il senatore Lumia afferma, e non è la prima volta che lo fa,

al semplice aderente all'associazione mafiosa di andare ad uccidere una persona. Quegli omicidi possono essere commessi solo solo l'ok da parte del vertice dell'associazione criminale, ma anche l'ok, quanto spontaneo non so, di chi comanda nel territorio in cui quell'omicidio deve essere commesso. Al senatore Lumia allora vorrei ricordare che questo tipo di atteggiamento, cioè l'ordinare, il consentire, il programmare un omicidio o un reato di pari gravità, per chi è al vertice di quella organizzazione, fa scattare la punibilità per il reato-fine ai sensi dell'articolo 110 del codice penale. Se il senatore Lumia dovesse avere la compiacenza di rinfrescare la sua memoria andando a leggere la sentenza del maxiprocesso 1 di Palermo o di tante altre sentenze, ad esempio del processo sulla guerra di mafia di Reggio Calabria o ai processi di Raffaele Cutolo, si troverebbe di fronte

e riteniamo che questo inasprimento sanzionatorio, attesi gli attuali tetti di pena, sia sostanzialmente inutile e non sia altro che un trabocchetto suggestivo che il Governo muove nei confronti della popolazione, del tutto similare a quello che sta accadendo per la corruzione, cioè è come se volesse dire «Vedete? Siamo arrivati noi, siamo durissimi nei confronti della associazione mafiosa», ma nella realtà quello che fa non porta risultato, perché qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è, ad esempio, tra l'attuale pena di 24 anni e la nuova, severissima pena che viene irrogata con questa legge, di 26 anni.

con l'articolo che si intende approvare e che è stato votato in Commissione si dice che l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i delitti previsti agli articoli 314 e 317, ossia tutti i reati contro la pubblica amministrazione, amministrazione, è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Il mio emendamento, condivide la *ratio* di questa norma, ma non la limitazione ai soli reati contro la pubblica amministrazione, non solo per un equilibrio sanzionatorio, ma essenzialmente per una parità di diritti tra i cittadini.

e che viene scippata davanti allo sportello della banca o dell'ufficio postale vedrà poi il ladro patteggiare e non restituire alcunché?

Una cosa è se affermiamo il principio secondo il quale chi chiede il patteggiamento deve restituire, se c'è un profitto,

all'articolo 3, ma qui invece venite a creare una disparità di trattamento. Il senatore Zanda non frequentava il dipartimento del Centro per la riforma dello Stato, all'epoca del terrorismo, quando Pecchioli correttamente invitava tutti all'equilibrio delle pene e a tener conto dei diritti della povera gente, di coloro che meno hanno e che hanno necessità di essere protetti. Questo articolo, invece, introduce una differenziazione senza tenere conto di coloro che meno hanno.

un qualsiasi guadagno illecito, deve restituirlo per essere ammesso al patteggiamento, è una cosa; ma limitarsi ai reati contro la pubblica amministrazione è incoerente e determina incostituzionalità per differenti trattamenti rispetto agli altri. Prendo atto che la maggioranza se ne frega di quelle che sono obiezioni di diritto, per la parità dei cittadini di fronte alla legge,

In cambio mi permetto di chiedere, solo per questo intervento, un minimo di attenzione all'Assemblea, considerando il fatto che, se è vero che ciascuno di noi vota

Personalmente ritengo che l'articolo 5, oggetto di questo emendamento, sia incostituzionale. So bene che la pregiudiziale di costituzionalità è stata già respinta dall'Aula, ma mi permetto, per quel poco di attenzione che intendete dedicarmi, di chiedere a voi per quale ragione questo tipo di patteggiamento condizionato non è richiesto per il corruttore, mentre lo è per il concusso indotto,

il corruttore generale, normale possa patteggiare senza la condizione, analoga cosa non possa fare chi commette lo stesso reato, per cui è prevista la stessa identica pena: in altri termini il corruttore dei membri della Corte penale internazionale, degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri. esteri. Dico questo perché nell'articolo 5 non vi è alcun richiamo al corruttore, non vi è alcun richiamo all'articolo 321 del codice penale,

che sarà oggetto dell'attenzione della Corte. Addirittura - ma questo è solo un elemento di colore - in questo articolo si prevede l'impossibilità del patteggiamento normale, quindi patteggiamento condizionato, anche per il reato di peculato d'uso, la cui pena è da uno a tre anni. Detto tutto questo sul piano della costituzionalità, vorrei fare con voi il seguente ragionamento: aderire aderire al patteggiamento significa la possibilità di ottenere una diminuzione della pena fino ad un terzo. Mi permetto di rammentare a tutti quanti voi che chiedere il giudizio abbreviato significa ottenere una diminuzione della pena secca di un terzo. Quindi, sotto il profilo della convenienza, è più conveniente il giudizio abbreviato rispetto al patteggiamento. È chiaro però che, patteggiandosi la pena,

dovrebbe accedere al patteggiamento con la restituzione del maltolto, quando la stessa identica strada sotto il profilo della pena può tranquillamente raggiungere con il giudizio abbreviato? E non vi è chi non veda e chi non sappia che il patteggiamento è utile non tanto ai fini della deflazione dei carichi giudiziari, quanto ai fini degli effetti che la sentenza di patteggiamento ha in tutti i procedimenti, i dibattimenti e quant'altro cui accedono i correi di chi ha patteggiato. Sotto questo profilo è estremamente emblematico quanto affermato proprio sul punto specifico dal procuratore aggiunto di Venezia Nordio, il quale, a chi si lamentava in ordine ad un tetto non particolarmente rilevante dei patteggiamenti, ha risposto di essere d'accordo e che forse noi abbiamo ragione, ma grazie a quei patteggiamenti l'accusa in dibattimento viene fortificata e, quando la gente comincia a patteggiare, iniziano a patteggiare tutti gli altri. altri. Siccome - per come vi ho detto - non vi è convenienza a percorrere il patteggiamento nelle condizioni date, perché gli stessi identici effetti - poco più o poco meno possono essere raggiunti con il giudizio abbreviato, credo che questo articolo sia profondamente sbagliato sotto il profilo costituzionale, ma principalmente anche sotto quello della pratica giudiziaria. E poi delle due l'una: se noi immaginiamo un patteggiamento condizionato per tutti i reati che prevedono un provento economico o qualche altra utilità, caso non vi è un problema di costituzionalità. Ma mi volete spiegare la ragione per la quale il concusso indotto deve patteggiare in termini condizionati e l'evasore fiscale no? no? Sbaglio o l'evasione fiscale è uno dei problemi prioritari e più importanti in questo Paese? E non ritenete voi che, nell'immaginare

del reato e quel provento o profitto del reato viene sequestrato nella fragranza del reato di corruzione, la restituzione è un di più rispetto al provento sequestrato? E come si muove sotto il profilo giuridico? Si muove come una riparazione pecuniaria, similarmente a quanto scritto nell'articolo 3, non potendo sicuramente essere un risarcimento del danno? Io ho l'impressione che anche qui

È vero che l'abbreviato determina la riduzione dell'intero terzo, laddove il patteggiamento determina una riduzione fino ad un terzo. Si tratta, però, chiaramente, di riti completamente diversi. diversi. Il patteggiamento determina la conclusione di quella vicenda giudiziaria in quella fase, ed è possibile soltanto per condanne fino a due anni di reclusione, fatta eccezione per il cosiddetto patteggiamento esteso, che non è neanche qui in discussione. Ovviamente c'è da osservare che l'abbreviato è possibile indipendentemente dai limiti

Il relatore si permette di dire che - come sempre accade - possono essere paragonate soltanto entità assimilabili, ma non entità talmente differenziate da determinare l'impossibilità di un raffronto che ubbidisca ai termini della razionalità. pone poi un problema nelle vesti della costituzionalità, per una asserita irragionevolezza e/o disparità di trattamento. La questione è certamente nota,

assolutamente ammissibile. Lo Stato prevede determinati istituti premiali e ne riduce l'applicazione con riferimento a situazioni

preveduti in via generalista per una serie di reati che sono preclusi, al contrario, per determinati reati. Non è mai stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale e credo che, se lo fosse stata, sarebbe stata rigettata, per la ovvia ragione che il principio di uguaglianza impone che situazioni identiche non possano essere trattate in maniera differenziata ovvero che situazioni differenziate non possano essere trattate in maniera identica. Ma, se situazioni differenziate sono trattate in maniera differenziata, non si pone in alcun modo il problema della violazione del principio di uguaglianza, nemmeno sul versante dell'articolo 3 e, quindi, del principio di ragionevolezza. salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «L. Calabrese-P. Levi» di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona,

con l'emendamento 6.300 si vuole introdurre un nuovo comma all'interno dell'articolo 165 del codice penale, che già conferisce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena

rispetto ai reati di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione presso organi delle Comunità europee ed altro. Si inserisce, per questi reati, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione e al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta, quindi, di un adempimento di natura pecuniaria necessario al riconoscimento del beneficio, che costituirebbe titolo di riparazione in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale (corruzione in atti giudiziari), in favore dell'amministrazione della È evidente che non stiamo parlando di risarcimento del danno, che ha altre finalità e rimarrebbe per questo impregiudicato. Stiamo parlando di una misura che ha l'obiettivo di intervenire in maniera più radicale

rispetto al profitto di un reato e, contemporaneamente, permette di ridurre il danno erariale subito dell'amministrazione pubblica. un'ipotesi in cui il reo non abbia la capacità economica di restituire quella somma e che, quindi, il risarcimento possa essere sostituito con la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

Sì, accetto la riformulazione. Rimane - immagino - valida la formulazione delle ultime due righe relative alla rubrica

e Lumia. Lo abbiamo già votato, relatore. L'articolo 3, che abbiamo votato, dice che con la sentenza di condanna per uno di questi delitti è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto da pubblico ufficiale

«Nei casi di condanna (...) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata». Ma come «la sospensione condizionale»? Se abbiamo votato che comunque la condanna,

qualunque condanna, anche nel limite della sospensione condizionale, porta già a questo risultato. Forse il relatore era distratto oppure è stato pressato dal collega Lumia e, quindi, ci siamo limitati solo alla seconda parte. Ma, in effetti, il testo è uguale a quello che abbiamo già votato e sarebbe ridicolo ridicolo prevedere l'obbligo di restituzione per la sospensione condizionale, quando anche un giorno di carcere, ossia qualsiasi sentenza di condanna, porta già quella conseguenza.

superfluo, che - come ben ha colto il senatore Caliendo - non serve veramente a nulla.

di ragionare e di far valere il diritto sancito dalla nostra Carta costituzionale. Non possiamo lasciare la parola solo a chi si intende di mafia, a chi si intende un po'

ben ha colto il senatore Caliendo. Stiamo facendo un emendamento fotocopia, che ovviamente serve solamente per propaganda e non certamente ai fini della giustizia.

non c'è dubbio che in questo caso si tratti di una materia speciale. Non stiamo dicendo che la condanna è subordinata a un qualcosa (l'evocazione dell'articolo 3). specifichiamo a cosa può subordinarsi la sospensione condizionale della pena. È chiaro, poi, che la sospensione condizionale della pena è un beneficio che si applica nei casi di condanna: se l'imputato è assolto, non gli deve essere sospesa la condanna, e questo mi pare di tutta evidenza. di una cosa già prevista nell'articolo 165 del codice penale, che disciplina, tra l'altro, le circostanze e gli adempimenti ai quali può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ora ripeto quanto ho detto all'inizio, dando conto

ma anche la riparazione, tant'è che, esordendo e dando conto del parere favorevole all'emendamento a prima firma del senatore Lo Giudice, io dissi che la ragione della soppressione condanna nei casi di patteggiamento, di cui all'articolo 3, oltre che con riferimento all'articolo 5, trovava giustificazione anche nell'emendamento 6.300, sul quale avrei espresso parere favorevole. quello che si perde sul versante dell'articolo 3 si recupera sul versante dell'emendamento 6.300, come avevo già detto all'inizio dell'illustrazione dei pareri.

e la società o la stazione appaltante non esegue e non si adegua all'ordine, cosa succede? L'Autorità anticorruzione dovrebbe rivolgersi al TAR o al giudice ordinario per ottenere l'eliminazione di quel provvedimento, quando saranno già finiti i lavori? Allora, con

che intervengono nella fase precedente all'effettuazione delle opere e volti, quindi, ad evitare qualsiasi ipotesi di corruzione attraverso una maggiore trasparenza ed una maggiore conoscenza da parte dell'Autorità anticorruzione

ad assumere un'iniziativa concreta. C'è un dato che risulta dalla presentazione del rapporto dell'organismo indipendente di valutazione sull'attività

obbligati a presentare la loro valutazione di trasparenza, tra cui 35 aziende sanitarie locali, 8 Autorità indipendenti, 20 Comuni Capoluogo di Regione, 13 Ministeri e 22 Regioni. Ebbene, cento dei Ministeri ha espletato tutte le procedure previste, pubblicando l'attestazione OIV (cioè quella relativa agli organismi indipendenti di valutazione), tranne il MISE, il Ministero dello sviluppo economico. Con questo ordine del giorno vorremmo che il Governo adottasse in maniera rapida tutte le opportune iniziative perché questa mancanza,

dell'occupazione delle istituzioni da parte del ceto politico per sistemare parenti, amici e amici degli amici e dispensare favori. Da noi è una prassi più che consolidata. Penso a tutti quei politici che nella scorsa legislatura sedevano in Parlamento o erano membri del Governo, ai quali dopo sono stati attribuiti incarichi in fondazioni, *authority*, enti ed organismi pubblici di vario tipo, talora di dubbia utilità, sia pure con le dovute differenze fra ruoli puramente formali e simbolici e posti di minore visibilità mediatica, ma di grande potere. Il problema ha trovato una soluzione solamente a livello locale, grazie ad un decreto nel 2013. Piena libertà, invece, per i pesci grossi (si fa per dire): chiunque abbia ricoperto ruoli nazionali (quindi ex Ministri, ex parlamentari ed ex Sottosegretari)

Ricordo che con questo emendamento si incide su un decreto attuativo della legge Severino, che ha trattato il tema dell'anticorruzione. Per questo ho presentato un solo emendamento al testo in discussione, che va proprio in questa direzione, precludendo il ricollocamento degli "ex" per due due anni dalla loro uscita dal Palazzo. Il Movimento 5 Stelle lo dice da sempre: la gestione amministrativa deve essere indipendente dai partiti. Basta inciuci, basta giochi di potere, basta favoritismi. questo emendamento potrebbe essere definito «norma anti-trombati». Io, più garbatamente, prendo in prestito le parole del presidente Renzi, 22 ottobre 2012, rivolgendosi a Giovanna Melandri, da poco nominata presidente della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, disse: «C'è una vita fuori dalla politica, c'è un mondo, la bellezza delle relazioni, mettersi in gioco nel privato, com'è possibile che ci sia ancora una via d'uscita come il MAXXI quando esci dal Parlamento?», e la definisco: «norma a tutela della bellezza delle relazioni». Invito tutti a votarla. Immagino che in particolare i colleghi del PD, prendendo spunto dalle parole del proprio segretario, non avranno problemi a dare il proprio sì.

La corruzione è dilagata, perché mafiosi e corrotti hanno un terreno comune: arricchirsi. «La corruzione in Italia è un fenomeno di sistema assolutamente dilagante, perché mai efficacemente contrastata e combattuta, ma anzi per troppo tempo tollerata e giustificata» e sul cui fronte vi è stato un «deciso arretramento quando sono state assicurate ampie prospettive di impunità per il falso in bilancio»; utilizzo e condivido queste parole del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Il Movimento 5 Stelle è stato sempre duro in materia di lotta alla corruzione e alla mafia e lo dimostriamo ogni giorno. Al momento, ci troviamo di fronte ad un sistema normativo insufficiente e contraddittorio e non mi riferisco solo alle pene per i delitti di corruzione di cui abbiamo più volte discusso: pensiamo, ad esempio, alla disciplina dell'inconferibilità degli incarichi amministrativi. Attualmente, il decreto legislativo n. 39 del 2013 individua i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, che comportano l'esercizio di funzioni amministrative e di amministrazione e gestione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, a soggetti interni o esterni alla pubblica amministrazione. Sono inconferibili, cioè è precluso il conferimento di incarichi, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale; coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. Da una prima lettura, emerge un'evidente contraddizione tra le cause ostative all'assunzione di incarichi amministrativi: non è contemplato il cosiddetto danno erariale, consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione, o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali, così come disposto dall'articolo 1223 del codice civile. Dunque, ricapitolando, se una persona cagiona un danno erariale e viene condannata a risarcire un ente pubblico per il danno cagionato, può continuare ad operare per lo stesso e continuare ad assumere altri incarichi, magari cagionando ulteriori danni in altre amministrazioni. Tutto questo non è accettabile, per questo motivo chiediamo al Governo, con quest'ordine del giorno, di primo è a provvedere alla revoca immediata di ogni incarico affidato dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici, da enti di diritto privato in controllo pubblico, a soggetti condannati - anche con sentenza non definitiva - per illeciti amministrativi, con particolare riferimento al danno erariale. Il secondo è a provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconferibilità degli incarichi amministrativi, anche per soggetti condannati con sentenza non definitiva, per illeciti amministrativi, con specifico riguardo

non tanto per chiedere che sia votato, quanto per evidenziare la stranezza delle norme e di come si interpreta l'anticorruzione da parte di questo Governo. L'articolo 7 ha previsto una serie di norme

approvata qualche mese fa dalle Camere è stata prevista una decurtazione di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione. Se questo è il modo di interpretare l'anticorruzione, se questo è il modo di interpretare l'aumento delle delle funzioni di un organo che oggi si sta rivelando importante e fondamentale nel denunciare e anche nell'esprimere pareri importanti sull'anticorruzione,

all'ANAC per gli anni 2015, 2016 e 2017. Invitiamo il Governo a ripristinare quei fondi togliendoli magari da qualche altro spreco.

dopo le parole "somme liquidate" inserire le seguenti: "le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2"». In questi termini di riformulazione

Stiamo parlando dei poteri di vigilanza dell'Autorità anticorruzione sulle pubbliche amministrazioni. L'articolo 1 della legge del 2012, alla lettera *f)*, prevede che l'Autorità eserciti la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5

«la Commissione» - cioè l'Autorità anticorruzione - «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5

La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati». Nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non adempia

trattandosi di pubblica amministrazione, l'Autorità anticorruzione possa adottare i provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e alle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza. Su questo emendamento viene però espresso parere contrario e non si capisce perché.

ma per i provvedimenti soppressivi di atti non ispirati alla trasparenza può solo limitarsi all'ordine, non può fare altro. La mia domanda è perché è stato

Do il riferimento normativo, se può essere utile per un riscontro: la norma che ha assegnato all'ANAC le funzioni della Commissione è quella disposta dal decreto-legge n. 101 del 2013, all'articolo 5,

Si tratta di individuare qual è l'autorità che ha la potestà di erogare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (il famoso decreto attuativo anche della legge Severino in tema di trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Stavamo chiarendo la ragione del parere contrario all'emendamento 7.302, perché ritenevamo che vi fosse una connessione con l'ordine del giorno G7.100, al quale si era dato parere favorevole. Peraltro, come questione di ordine generale, perché altrimenti non si capiscono le ragioni del sì e del no, si era ripetutamente detto in Commissione anche nel corso dei lavori che le norme di natura preventiva sono assolutamente necessarie che mancava, nel contesto del dibattito, un documento razionalmente orientato e completo in materia di prevenzione. Il testo sulla prevenzione deve essere un testo organico. La Commissione ha ritenuto di non potere intervenire in maniera estemporanea sul tema della prevenzione, perché questo tema deve essere oggetto di un testo complessivo. Noi non possiamo intervenire di volta in volta, tant'è che i pareri favorevoli sono mirati agli obblighi informativi, per allargare l'informazione.

Grazie

si legge che gli incarichi di studio e gli arbitrati sono forme spurie adottate dalle pubbliche amministrazioni per la corruttela.

tutta una serie di principi che ho visto i colleghi hanno presentato separatamente negli emendamenti successivi. Presentando questo emendamento faccio anche una sorta di dichiarazione rispetto alle tracce, che saranno accolte o non accolte, presenti negli emendamenti successivi. In buona sostanza, quello che succede con il falso in bilancio*...

quest'Aula, rispetto al quale tutti si vogliono appuntare delle stellette sul petto, quindi forse sarebbe il caso che capissimo sia cosa stiamo facendo sia cosa non stiamo facendo.

che è «un ingiusto profitto» per sé o per altri. Di fatto questa è una limitazione della portata applicativa; è infatti difficile dimostrare che l'attività sia stata compiuta

fingere che un'attività sia ancora in buona salute, quando magari è completamente decotta. Si potrebbe dire che questo è un ingiusto profitto indiretto; però, di fatto, possiamo anche dire che a volte non c'è un ritorno per i soggetti che siano autori del reato stesso o per qualcun altro. Rimane comunque il fatto che si tratta di un grave danno che viene procurato a chi con quella società ha oppure ha avuto rapporti.

al posto di «informazioni», perché l'espressione «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» esclude tutta la parte relativa alle valutazioni, che tra l'altro spettano proprio ai vertici, nel momento in cui si forma il bilancio.

avrò un valore totale di 1 milione di euro. È chiaro che il fatto materiale consisterebbe nel modificare il numero dei veicoli che ho in magazzino; dei veicoli stessi, comunico comunque un'informazione falsa, ma non un fatto materiale non rispondente al vero, perché si rimane nell'ambito delle valutazioni.

di applicare questa norma, perché occorre che ci sia una condotta decettiva e, allo stesso tempo, questa condotta deve esserlo in concreto. Tra l'altro, non si risolve il problema

con l'articolo 8 si fa un passo in avanti, perché si reintroduce il principio della punibilità del falso documentale societario e si consente alla giurisdizione di tornare a tutelare gli interessi dei creditori e dei risparmiatori. Però ci sono troppi paletti e troppe trappole. Si distingue tra l'ambito delle società non quotate e quello delle quotate e questo può essere ragionevole. La condotta incriminata è l'esposizione di fatti non rispondenti al vero e questo non mi preoccupa perché tutti i fatti sono, in qualche misura, oggetto di valutazione, posta più, posta meno. Una stima può essere palesemente falsa se totalmente sganciata dai valori contenuti, ma il testo proposto forgia un reato a dolo specifico con una tale scalettatura che sembra fatta apposta per gli azzeccagarbugli berlusconiani. Si mette il falso commissivo e quello omissivo; c'è quello nelle società quotate e quello delle società non quotate. Poi c'è la necessità che il falso sia idoneo concretamente a indurre il lettore in errore.

che non basta: è prevista una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e un'ipotesi scriminante per quelli di particolare tenuità. Allora, mi domando e dico: a che serve quel termine «rilevanti»? C'è un limite di finalità; c'è l'idoneità della condotta; ci sono le ipotesi attenuanti attenuanti e quella scriminante. A che serve dire che il solo falso punibile è quello sostanzioso o rilevante? Oltre che sul piano logico, quella parola è anche una sgrammaticatura giuridica.

agroalimentare di Treviso. Insomma, la rilevanza è un concetto del tutto indeterminato e contrastante con l'articolo 25 della Costituzione. Invito, quindi, ad approvare l'emendamento 8.311, che, peraltro, va incontro ai rilievi espressi nel parere della Commissione affari costituzionali.

Signora Presidente, vorrei ricordare a tutti che da sempre nel falso in bilancio, quando si parla di comunicazioni non rispondenti al vero, è sempre stata aggiunta la frase

Vorrei ricordarvi un articolo sul «Corriere della Sera», a firma di Ferrarella, il quale dice che dal testo sono state espunte le valutazioni. Per cui, a una lettura letterale, il testo porta ad escludere che le valutazioni possano rientrare nel reato. Rispetto a questa incongruenza e indecisione o genericità della norma, come volete chiamarla, vi chiedo di valutare quale può essere la posizione di un'azienda straniera che deve venire a investire in Italia. Prima di investire, ovviamente vuole rendersi conto di quale sono le norme penali che sovrintendono alla corretta gestione delle informazioni sociali. Nell'ipotesi di specie, la domanda è la seguente: se voi vi trovaste al posto dell'amministratore delegato di quella società,

che un determinato fatto, che io devo comunicare dipenda da stime e che, per ipotesi, i miei esperti e consulenti a cui mi sono rivolto siano quattro commercialisti

Vogliamo affossare definitivamente l'economia italiana già in crisi? Vogliamo mettere le piccole imprese nell'impossibilità di funzionare? Liberi di farlo. Per il momento, signora Presidente, mi limito a dire che comunque questa precisazione è necessaria all'interno del testo.

nell'intervento che ho fatto allorquando ho commentato gli emendamenti, ci sono tutte le risposte alle questioni che sono state poste. Nessuno ha la presunzione di dire che la propria risposta è la verità, dal punto di vista della completezza delle argomentazioni, ognuna delle obiezioni che sono state proposte in questa sede ha già avuto, in due occasioni, un'articolata risposta. Siccome, però, è giusto che il dibattito sia il più possibile approfondito e articolato e che le questioni, ancorché trattate, lo siano ulteriormente, visto che gli argomenti usati non hanno avuto l'efficacia persuasiva di indurre a diverse considerazioni, è giusto che il relatore si spenda ulteriormente. La prima delle questioni proposte fatti rilevanti. Io ho reiteratamente detto che l'espressione «rilevanti», l'aggettivo «rilevanti», non è usato come elemento quantitativo indeterminato. in questo caso si potrebbero porre quei problemi di costituzionalità in relazione alla sentenza del 1989, n. 247, della Corte costituzionale. Io uso il condizionale («si potrebbero porre») vero che quella sentenza sia generalizzante. Quella sentenza dice con assoluta chiarezza che non è possibile che l'intero carico di disvalore di una fattispecie graviti su elementi indeterminati di tipo quantitativo della fattispecie, perché, se questo carico di disvalore gravasse su elementi della condotta,

relatore. Colleghi, credo che il relatore stia facendo uno sforzo per rispondere alle obiezioni che sono state sollevate su un tema molto delicato; quindi, vi pregherei di abbassare il tono della voce

di tutte quelle componenti dimostrative di una evidente pregnanza fattuale della componente oggettiva come del suo versante soggettivo. Voglio dire che il fatto è un fatto iperdeterminato e che l'attributo di rilevanza

è libero di poter dire che queste spiegazioni non convincono; nessuno ha la pretesa di convincere gli altri - ma adesso lo faccio per la terza volta: «rilevante» significa un fatto materiale dotato di una capacità concretamente offensiva dell'interesse giuridicamente protetto. Questo lo si fa nel solco di una giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce il principio di offensività in due dimensioni tra di loro concorrenti: in senso astratto, perché la norma deve essere popolata di elementi dimostrativi della astratta offensività della condotta; in senso concreto, perché questo richiamo richiamo contenuto nel testo della norma impone al giudice una interpretazione che noi qualifichiamo come orientata all'offesa. Quindi, rilevante vuol dire offensivo dell'interesse giuridicamente protetto, ovviamente nel solco di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. D'altronde, come ho già detto - e mi permetto di invitare i colleghi senatori a riflettere, poi certamente a dissentire «rilevante» è attributo non di un elemento quantitativo. Qui nessuno ha scritto variazioni, entità, quantità rilevanti; qui si è scritto «fatti materiali rilevanti» e il principio di materialità, evocato con assoluta chiarezza dall'attributo «materiali», è connesso ai fatti, e quindi a dimensioni ontologiche e non a categorie dello spirito. Quando si parla di fatti si indica una realtà ontologica, una circostanza che è dotata di una sua materialità, per l'appunto; si evoca un principio, quello di materialità, che storicamente è connesso nel diritto penale alla offensività. Quindi, noi diciamo, per ben tre volte, che ci deve essere un fatto, quindi un'entità dotata di consistenza ontologica; questo fatto deve essere materiale, e che per di più deve essere un fatto offensivo. Allora non si può dire che questa è una condotta indeterminata. Qui non stiamo parlando di alcunché che riguarda l'evento perché sono reati di pura condotta, tra l'altro costruiti sul pericolo; l'evento è una circostanza possibile, ma non necessaria al fine della sussistenza degli elementi del tipo legale. contro il dolo specifico, dicendo che è difficile provarlo. Queste sono affermazioni che vanno sfatate una volta per tutte. Dei problemi probatori non si può far carico certamente il legislatore, ci mancherebbe altro: il problema probatorio è un problema che dà serietà e consistenza, senatrice Mussini, alla norma penale ed incriminatrice, perché le conferisce le conferisce quel requisito di concretezza che impone agli organi titolari dell'azione penale di dimostrare le peculiarità e le specificità della norma penale incriminatrice. Dire poi che sono elementi difficili da provare significa ignorare che il furto è costruito sul dolo specifico, altrimenti non avremmo mai potuto condannare nessuno per furto perché c'è scritto «al fine di trarre profitto». Sono cose di una tale evidenza che il relatore

questo fa parte della grammatica giuridica, non è necessario intervenire addirittura davanti al Senato per spiegare che «altri» significa persone diverse dall'autore del fatto, tant'è che la legge dice, proponendo una opposizione

peraltro, è un'espressione che sta nel codice dal 1930 e non possiamo meravigliarci di espressioni collaudate da 85 anni di applicazione del diritto penale, perché costituisce ovviamente un vero e proprio paradosso. all'ingiusto profitto, anche qui francamente potrei esimermi dal dire che questa espressione sta nel codice penale da sempre, chiaramente per quei reati rispetto ai quali il legislatore, nell'ambito di una discrezionalità che non gli può essere negata (se (se c'è qualcuno che pensa che le norme penali si scrivano con il *computer* mi permetto di dire che non è così) non segue delle categoria preontiche che gli impongano da una parte o dall'altra di orientarsi per come taluno pretende che il legislatore si debba orientare. Il legislatore fa delle scelte, peraltro il dolo specifico significa mirare ad un fine, la realizzazione del quale non è richiesta ai fini della sussistenza del fatto di reato, quindi è sufficiente dimostrare che taluno abbia agito ad un fine, ma poi quel fine non è necessario che si sia realizzato perché il reato sia punibile. Tant'è che noi diciamo che il dolo specifico è un arretramento del momento della punibilità, finisce per determinare un allargamento del campo di applicazione della norma penale incriminatrice. che in una perdita di bilancio non c'è un profitto è una cosa che francamente non riesco a capire, perché è chiaro che l'occultamento di una perdita determini un vantaggio per il soggetto che si avvale di questa mistificazione, di questo nascondimento: se una perdita non la si porta in bilancio, questo è un vantaggio. È chiaro che i concetti non sono antitetici, ma anzi perfettamente consonanti l'uno rispetto all'altro. Ci si lamenta di questi diversi livelli. Le norme - mi sia consentito - vanno interpretate e capite e quanto all'interpretazione, approfitto per anticipare un concetto: nessuno può pensare che noi oggi in Senato

Noi riteniamo di avere scritto, e di avere prima ancora pensato, delle norme ragionevoli e conformi ai nostri principi. Ovviamente dobbiamo, come in ogni caso del genere, prefigurare che ci saranno dei tribunali, delle corti d'appello una Corte di cassazione le quali poi daranno risposta ai nostri dubbi. A noi basta aver scritto delle norme che si inseriscono in un quadro di natura costituzionale. Bene, noi abbiamo fatto un fatto base, un fatto materiale offensivo. Rispetto a questo fatto, in via scalare e subordinata, come valore successivo in un ordine gerarchico che vede al primo posto inserita la categoria dei fatti materiali rilevanti, abbiamo i fatti di lieve entità. Illustri senatori, i fatti di lieve entità stanno nel sistema penale da sempre. Noi abbiamo addirittura la possibilità di dire che l'elemento indeterminato, allorquando faccia parte di una norma favorevole, non pone alcun problema di legittimità costituzionale,

Caliendo ha posto ripetutamente questo problema: insomma, le valutazioni stanno o non stanno dentro i fatti materiali rilevanti? Qui non do la mia interpretazione, non perché non abbia una risposta (perché io una risposta ma non credo che il relatore debba dare una sua interpretazione. Questo è un problema interpretativo e qui non c'è da scandalizzarsi, perché sappiamo bene che i giudici interpretano le norme. Il relatore è convinto di quello che dice...

possano o meno rientrare all'interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti. Ripeto, il relatore a tal proposito non dà alcuna risposta, perché non la deve dare; ci mancherebbe altro che la desse. Noi non siamo la Corte di cassazione che dà risposte giurisprudenziali; questo è un tema che la giurisprudenza affronterà. Ripeto, il relatore ha la sua risposta, la sua risposta, ma non avrebbe alcuna efficacia e alcun significato vincolante, pertanto il relatore ritiene non di non poterla dare, bensì di non dover dare alcuna risposta su questo aspetto. "Consapevolmente": l'ho anche detto: l'avverbio «consapevolmente» ha una doppia funzione: la funzione di... *(Brusio)*. Signora Presidente, il relatore parla anche per ore, però è un paradosso che taluni si lamentino

che l'impostazione della questione trattata dagli articoli 8 e 9 sia stata avviata, e mi risulta che ci sia un'intesa sostanziale dei Gruppi per riprendere la discussione del provvedimento domani mattina,

come un vero sistema che si sviluppa intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo e lavorazione di prodotti forestali,

Oltre alla produzione, è presente anche un magazzino prodotti finiti automatizzato tra i più grandi esistenti: 6.000 metri quadrati con una capacità di 32.000 tonnellate di carta. Adesso nello stabilimento di Verzuolo l'azienda ha intenzione di aprire unilateralmente la procedura per il licenziamento collettivo di 46 operai e lo ha comunicato ieri alle rappresentanze sindacali presso la sede Confindustria di Cuneo, come conseguenza dell'annunciata modifica dell'orario di lavoro su una delle due linee produttive giudicata maggiormente in sofferenza dalla proprietà. Nella storica cartiera a partire dal 2008 è stata avviata una riorganizzazione che, d'intesa con i sindacati, ha portato alla riduzione alla riduzione di circa 100 posti di lavoro per arrivare all'attuale forza produttiva di 400 dipendenti;

*(PD)*. Senza accordi tra proprietà e sindacati il rischio è di dare inizio a una serie di tensioni che porteranno scarsi risultati, con l'irrigidimento delle parti in campo a scapito di un accordo che, come è accaduto nel recente passato, possa essere occasione di presidio e rilancio dello stabilimento, consentendo anche all'azienda di ottimizzare i costi. Ho depositato oggi un'interrogazione ai Ministeri dei lavoro e dello sviluppo economico per sollecitare un loro intervento. Questa situazione rischia di portare tensioni e incertezze sul territorio del saluzzese, nell'area della Provincia di Cuneo, in cui è ubicato lo stabilimento di Verzuolo. Teniamo conto che sempre la Burgo solo sei mesi fa ha chiuso lo stabilimento di Cuneo della Comecart, azienda del gruppo specializzata in produzione di macchinari e componenti per l'industria della carta e officina di riferimento per le cartiere Burgo, mettendo in mobilità per cessazione di attività ben 39 dipendenti.

in questo caso non le ha revocate solo nel caso in cui Masciari si trovi in Calabria. Nel 1992 Pino Masciari si ribella alla 'ndrangheta, subendo gravi ripercussioni in ambito lavorativo e familiare, cominciando ad essere oggetto di furti, incendi, danneggiamenti e minacce. Alcuni malavitosi avvicinarono uno dei suoi fratelli e gli spararono alle gambe. Pino, che nel frattempo aveva subito numerose perdite economiche, fu costretto dai malavitosi a non costituirsi parte civile. che ha contribuito ad assicurare alla giustizia molti malviventi, non abita più in Calabria da anni, ma questa non è una motivazione sufficiente. La 'ndrangheta è dappertutto e le ultime vicende ancora una volta ce lo dimostrano. Oggi, lo Stato abbandona chi si espone per denunciare il malaffare, le ritorsioni, il sistema mafioso che sempre di più opprime i liberi cittadini del nostro Paese. Come possono gli italiani fidarsi di uno Stato che chiede ai suoi cittadini di denunciare il malaffare e poi, quando il cittadino è minacciato, lo abbandona? Spero si tratti solo di una incomprensione, altrimenti verrebbe da pensare veramente a qualcosa di drammatico e pericoloso per quella che continuiamo a chiamare Italia. Non possiamo che unirci agli appelli e alle petizioni che numerosi cittadini, e svariati consigli comunali e regionali

Signora Presidente, mi rivolgo a lei, ma il mio intervento è indirizzato all'Aula intera. Dalle notizie di stampa di questi giorni apprendiamo che il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone ha chiesto alla Sogesid di valutare l'adozione di un provvedimento in autotutela al fine di revocare l'aggiudicazione all'associazione temporanea di imprese TreErre/Italrecuperi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori dei messa in sicurezza della discarica Resit di Giugliano in provincia di Napoli. SpA è stata, infatti, giudicata inidonea ad eseguire i lavori per l'invaso che appartenne a Cipriano Chianese, il re delle ecomafie. risulta tra le aziende coinvolte nelle false bonifiche di Bagnoli e alcuni suoi membri risultano nell'inchiesta di mafia capitale. Come è potuto accadere ancora una volta che appalti siano stati affidati senza controlli? Era il 5 febbraio 2014 quando in quest'Aula, in sede di approvazione del provvedimento sulla cosiddetta terra dei fuochi, per l'ennesima volta non siamo stati ascoltati; anzi siamo stati derisi. Avevo personalmente chiesto di eliminare l'emendamento introdotto alla Camera che permetteva di andare in deroga alle norme in materia di antimafia per gli appalti delle bonifiche nella terra dei fuochi: sarebbe stata una pazzia e si sarebbe tradotto in un appoggio a norma di legge alla criminalità organizzata. Ci fu detto che non sapevamo leggere e che andare in deroga significava migliorare la norma. Sì, lo so, suona ridicolo, ma questa è stata la risposta della maggioranza. Signora Presidente, è successo. Già nel mese di gennaio, prima dell'approvazione del provvedimento sulla terra dei fuochi, c'erano stati i primi casi di aziende legate al *clan* dei casalesi che avevano provato a mettere le mani sul primo bando di gara delle bonifiche, in particolare sempre sulla discarica Resit. Eppure, nonostante i fatti noti e da noi denunciati in quest'Aula, l'emendamento si è trasformando in legge ed oggi, come al solito, a pagarne il prezzo sono i cittadini. Visto che si sta giocando con la vita delle persone e visto che il Movimento 5 Stelle aveva avuto ed ha ragione da vendere, gradiremmo almeno le scuse, che non sarebbero dirette a noi, ma ai cittadini che nella terra dei fuochi stanno morendo ogni giorno. sicurezza continua ad allarmare sempre di più, ma purtroppo altri episodi ci dicono quanto il Governo stia sottovalutando le circostanze. Proprio la scorsa settimana a Varese nel centro nel centro della città, in via delle Medaglie d'Oro, è accaduta una vicenda a dir poco paradossale e drammatica. A un posto di controllo 30 stranieri clandestini extracomunitari hanno circondato gli agenti di polizia, i quali hanno avuto la peggio. Il fatto è stato riportato dalla cronaca locale ha allarmato molto i cittadini, ma ancora di più gli agenti delle Forze dell'ordine. «Non siamo tutelati. Non abbiamo mezzi. Chiunque si sente in diritto di poterci accusare o aggredire. Ma noi non siamo né picchiatori né violenti. Siamo persone normali,

soffocata dall'aggressione di persone che nulla hanno a che fare con il nostro contesto di vivere civile e che, unite assieme in branco, si fanno forza e aggrediscono, anche le Forze dell'ordine, e mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

faccia un giro in piazza, si confronti con questa realtà e si renda conto che lasciare le Forze dell'ordine senza gli strumenti normativi e, ancora di più, i cittadini senza la garanzia che lo Stato reprima queste situazioni significa lasciare il Paese allo sbando. Noi su questo siamo molto arrabbiati. Sono sicura che il sottosegretario Pizzetti trasmetterà al Ministro dell'interno l'invito del senatore Candiani.

Grazie